L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio,

alle ore 14, presso la sede di palazzo San Macuto per procedere alla propria costituzione. **Informativa reca: «Informativa del Ministro del turismo sui fatti connessi a un servizio giornalistico televisivo e successivi articoli di stampa».

spero vorrete darmi atto che, a fronte della richiesta di alcuni Gruppi di opposizione - e sottolineo: alcuni e non tutti ho subito dato la mia disponibilità a riferire in Senato su una vicenda per la quale qualcuno, anzi, considera addirittura eccessiva questa mia decisione. Ma ho preferito non far pesare al Governo e alla maggioranza di cui faccio parte le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti. Ieri - come potete immaginare - ho riordinato le idee ed ho preparato una scaletta di quanto, in piena sincerità, oggi a tutti voi avrei dovuto illustrare. devo, però, dire la verità: stamattina è accaduto qualcosa che va veramente oltre la mia vicenda e che credo dovrebbe allarmare tutti voi, senza distinzione di appartenenza partitica o politica. Affermo, innanzitutto, sul mio onore, che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che, anzi, per scrupolo, ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi in proposito. E così mi è stato confermato. Ho anche estratto il certificato dei carichi pendenti, in cui risulta che non ci sono annotazioni per qualsivoglia procedimento nei miei confronti. Ripeto che stamattina un quotidiano, segnatamente il «Domani», afferma con dovizia di particolare che invece sarei indagata, sia pure segretamente, e snocciola informazioni, mescolando dati noti e altri oscuri, senza minimamente indicare alcuna fonte. Ebbene, delle due l'una: o questo giornale mente, sapendo di mentire, e sceglie proprio questo giorno, il giorno del mio intervento in Aula, per quella che si definisce una classica imboscata, non importa quanto veritiera, per colpire proditoriamente un Ministro del Governo contro cui giornalmente si scaglia; oppure prendo anche in considerazione una ipotesi che va a ripetere in piccolo vicende - ahimè passate della storia della politica italiana. Il «Domani» ha avuto una notizia che io - lo sottolineo - non ho e che nessuno potrebbe lecitamente avere. Sarebbe questa un'ipotesi ancora più grave della prima, tale - io credo - da mettere in subordine quanto ho in animo di illustrarvi e da rendere invece necessaria una comune azione del Senato contro - lasciatemelo dire queste sporche, schifose pratiche, contro quelli che si definiscono attacchi vergognosi, calibrati nel tempo e nei modi per rendere impossibile una risposta puntuale. Il «Domani» vuole alzare l'asticella, quando stanno invece per cadere le incredibili accuse dei giorni precedenti. Vi chiedo accoratamente di reagire a una tale pratica che oggi tocca a me e domani potrebbe colpire qualsiasi cittadino, politico o non politico. Esporrò comunque tutte le informazioni che mi avete richiesto e dopo aver precisato che, se avessi ricevuto un mai arrivato avviso di garanzia, ve lo avrei detto, perché per me non sarebbe cambiato nulla; non sarebbe cambiato di una virgola quanto sto per dirvi, né la mia fiducia nella magistratura, né tantomeno le mie convinzioni sulla mia vicenda, che - piaccia o non piaccia - non è tale da poter accontentare chi chiede quotidianamente le mie dimissioni. Oggi, più che darvi risposte, dovrei chiedere a voi con forza delle risposte dopo aver letto il «Domani» questa mattina. Qualcuno dovrebbe dare a me delle risposte. Possiamo stare tranquilli, perché abbiamo tutto il tempo. Io rispondo a qualsiasi domanda. Non vi fate prendere dai nervosismi. PRESIDENTE. Prosegua, Ministro. GARNERO quindi, che avrei bisogno di avere risposte e le chiedo con forza e vi chiedo: ma è normale che un Ministro della Repubblica, mentre sta per rivolgersi ai senatori, legga che secondo un giornale sarebbe indagato? Vi chiedo: è un Paese normale quello in cui un giornalista può scrivere che conosce cose a suo dire segretate dalla magistratura e ignote all'interessato e ai suoi avvocati che lo escludono? È normale? Certo, forse il giornale stamattina avrà - mi auguro - venduto qualche copia in più; forse chi temeva il mio chiarimento in Aula si potrà pure rallegrare di questa manovra e di queste notizie. Ma voi lascerete che tutto questo accada impunemente? O ci scandalizzeremo per come mi vesto, per dove abito, per le mie case, per come conduco le mie aziende, per i nomignoli che negli anni mi sono stati appioppati o per le mie amicizie? O chiuderemo tutti e due gli occhi su questa sporca pratica? Lo chiedo semplicemente alla vostra coscienza, se non fosse per il rispetto che io porto per quest'Aula, dopo l'uscita proditoria del quotidiano «Domani» chiuderei qua il mio intervento. Ma, aspettandomi un segno concreto di reazione da parte di tutti i colleghi, mi faccio forza e provo a riprendere il filo dell'intervento che avevo in animo di illustrarvi. illustrarvi. Voglio chiarire di essere qui non per rispondere a trasmissioni televisive o articoli scandalistici, ma per bloccare la strumentalizzazione politica che da settimane si sta facendo contro di me attraverso mistificazione della realtà. Sono qui principalmente perché voglio difendere il mio onore e, se mi consentite, anche quello di mio figlio,

Ci tengo però a precisare che risponderò vestendo i panni dell'imprenditore, perché è in tale veste che sono stata pretestuosamente presa di mira per indebolire la solidità e l'armonia con cui sta operando il Governo sin dal momento del suo insediamento. Del mio operato come Ministro posso semmai, forse, vantarmi del giudizio estremamente positivo che hanno espresso - bontà loro - anche in questi giorni i colleghi Ministri e lo stesso Presidente del Consiglio. E di questo voglio ringraziare tutti. Vi parlo quindi da imprenditore.

con quella passione che caratterizza tutti gli imprenditori, con la forza del lavoro, senza capitali di famiglia, contando solo su me stessa. In questi anni ho raccolto importanti successi imprenditoriali di cui vado orgogliosa e sono anche fiera di aver dato lavoro a tante persone. Tra le varie attività che ho portato avanti in oltre trent'anni, negli anni '90 ho creato e gestito una società che in pochi anni si è affermata sul mercato delle pubbliche relazioni nell'organizzazione di eventi.

io ho avuto il coraggio, come molti, di intraprendere molteplici imprese nella mia vita e poi sicuramente chi fa può sbagliare. Sono entrata nel settore dell'editoria appena prima che iniziasse la crisi mondiale della carta stampata. Sapete bene tutti quante testate hanno chiuso in tutto il mondo in questi anni: non devo venire a raccontarvelo io oggi. Il declino dell'editoria ha colpito anche l'attività della raccolta pubblicitaria e questo lo sappiamo. Poi sono arrivati quello che non vorrei stare qua a raccontare, il Covid, e quindi l'aumento dei costi della carta. Ma credo che tutti quelli che oggi in Italia fanno impresa possono capire molto bene quello che sto dicendo, perché anche loro si sono rimboccati le maniche, hanno lottato e stanno lottando per tenere in piedi le imprese - come avevo fatto io - specie in quei settori nei quali la crisi è stata più forte e globale. Anche le mie imprese di pubblicità e dell'editoria hanno subìto le conseguenze di tali crisi e da tempo - come vi ho detto - sto lavorando con tutte le mie forze, mettendo in gioco - e ne sono fiera, non me ne vergogno - l'intero mio patrimonio personale, perché credo nelle cose che faccio. Non mi sono mai nascosta

per cercare di uscire dalla crisi com'è giusto fare, ma sono qui per dire che non mi sono mai appropriata di nulla che non mi appartenesse, che non ho mai abusato delle mie posizioni apicali nelle aziende sfido chiunque a dimostrare il contrario. Sono qui però soprattutto per tentare di far comprendere - in ballo, lo ripeto e lo sottolineo, c'è il mio onore che i pretesi scandali esplosi nelle ultime settimane sono il maldestro tentativo di impedire alle aziende che ho fondato di portare a compimento la ristrutturazione in corso, facendo legittimamente ricorso agli strumenti messi a disposizione di tutte le imprese dai precedenti Governi e che sono ancora tuttora vigenti.

Ciononostante, vi assicuro che il mio progetto di ristrutturazione è molto più virtuoso di altre aziende nelle stesse condizioni. Essere un imprenditore e anche un politico non può voler dire che possa essere inibito il ricorso alle leggi vigenti per tutti: alcun favoritismo, assolutamente alcuno, ma nemmeno un'indebita penalizzazione *ad personam.* Non basta che io possa essere percepita come un simbolo di ciò che sicuramente non piace alla sinistra o che magari non piace nemmeno a qualche giornale, ma ciò non può permettere che io sia privata di quei diritti che sono riconosciuti a tutti. che la persona a cui attingono i miei detrattori come grande accusatore, a differenza di quello che è stato riferito da trasmissioni televisive, da siti, *blog* e dai giornali, non è un piccolo risparmiatore che lotta contro il capitale. Ma - secondo le notizie che lui stesso ha divulgato - è una sorta di finanziere che è partito molti anni addietro da Torre del Greco, si è trasferito prima a Londra, poi in Svizzera e successivamente a Montecarlo e ora risiede alle Bahamas. Non mi pare proprio il più titolato a ergersi ad accusatore di chi secondo lui non vorrebbe pagare le tasse allo Stato italiano.

ad accordi per me inaccettabili. Questo, però, è un tema a parte su cui purtroppo non posso aggiungere altro, perché sarà oggetto di apposita inchiesta giudiziaria che chiarirà, anche grazie a registrazioni vocali, le finalità che hanno ispirato chi ha attivato tutto ciò. Venendo ai chiarimenti in relazione a specifici fatti che mi sono stati contestati da giornalisti televisivi e dalla carta stampata, desidero precisare alcuni dettagli del tutto omessi, anzi artefatti nella trasmissione televisiva da cui tutto ciò è partito e che aveva uno scopo, sì: quello di creare collegamenti inesistenti, dubbi malevoli e odiosi sospetti. Non ho mai avuto il controllo o partecipazione di un qualunque rilievo nelle imprese del settore dell'alimentare biologico e della sua distribuzione, come molti *media* hanno raccontato per ben due settimane. Lo ripeto: mai. In realtà, ho svolto attività d'impresa nel mondo della pubblicità, dell'intrattenimento e dell'editoria. Venendo al punto, la mia partecipazione in Ki Group Srl, di cui alcune televisioni e testate giornalistiche hanno parlato diffusamente,

Un'altra notizia: nel 2010 il salvataggio di questo gruppo del settore biologico, che avviene dal *crack* Burani, è stato fatto o pensato non da me, ma dal padre di mio figlio, con cui già all'epoca non avevo più alcuna relazione affettiva e tanto meno di convivenza. Tra l'altro, il suo investimento in questo settore, ad onore del vero, ha fatto sì che i dipendenti del gruppo avessero davanti a sé anni di attività lavorativa remunerata, visto che ha acquistato l'azienda da un concordato preventivo, peraltro creando per un periodo un importante valore in borsa del gruppo, da zero, non dissipandolo. Grazie all'operazione di salvataggio in questione, quel gruppo aveva raggiunto un valore multimilionario in borsa. Dunque - ripeto - quel valore è stato creato da zero e non distrutto, al contrario di quanto sostengono alcuni. Quello che però è più importante ai nostri fini è che io non ho avuto alcun ruolo né nella sua fortunata costruzione né nel suo abbattimento. Spero di essere stata chiara. In ogni caso, non posso e non intendo rispondere delle scelte imprenditoriali del padre di mio figlio né posso raccontarvi - ne sono estranea e voglio rimanere e non voglio occuparmi di come proseguirà la sua storia imprenditoriale. Comunque, voglio essere del tutto trasparente: da gennaio del 2019, per meno di due anni, ho assunto una carica sociale in Ki Group Srl senza alcun potere operativo. Da allora sono cessata da tutte le cariche sociali in tale gruppo e ho messo una cesura totale con loro dopo che già un anno prima ero rimasta proforma nel consiglio. Con riferimento invece ai compensi milionari che mi sono stati attribuiti, vorrei precisare quanto segue: da Ki Group Srl negli anni 2019, 2020 e 2021 ho incassato complessivamente 27.000 euro lordi, in tutti e tre gli anni, con una media di 9.000 euro all'anno. Per gli anni precedenti 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, anni in cui la Ki Group Spa ha fatto margini operativi sempre largamente positivi, ho percepito dalla capogruppo mediamente un valore lordo annuo di circa 100.000 euro in maniera fortemente decrescente negli ultimi tre anni. Anche questa notizia era perfettamente a conoscenza di chi ha omesso di riferirla e si è invece limitato a fornire l'importo di compensi stratosferici molto diversi da quelli che io ho preso. Così come era perfettamente noto che gli stipendi e il TFR di Ki Group, ancora da corrispondere ai dipendenti, erano inerenti al personale fuoriuscito dall'azienda nel corso dell'anno 2023, quando io già da tempo non avevo alcun ruolo. Tuttavia, per potervi rispondere precisamente, ho chiesto informazioni e posso comunicarvi che i lavoratori dipendenti della Ki Group Srl verranno integralmente soddisfatti con riguardo a tutti i loro diritti di credito. Questo lo potete verificare perché è scritto nell'accordo di concordato. Poiché infine sono stata chiamata a rispondere riguardo a questo gruppo che non ho mai gestito, faccio una doverosa precisazione su un tema specifico: la società, nell'immediato seguito dell'emergenza Covid, fece richiesta di accesso, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, a un prestito obbligazionario erogato da Invitalia. Poiché l'erogazione di quel prestito era subordinato a un impegno alla capitalizzazione anche da parte dei soci, quale socia, pur di ampia minoranza (5 per cento), ho fatto ovviamente la mia parte e, se vi fa piacere, posso dirvi che ho anche perso tutto l'investimento che avevo intrapreso. Questo l'ho fatto perché ha coinciso con l'ingresso di mio figlio, andato a lavorare con il padre. È ovvio che in casa - e non credo sia vietato dalla legge - mi poteva parlare e mi ha parlato delle difficoltà che incontrava. invece arrivare al mio gruppo, quello che orgogliosamente ho fondato e di cui mi assumo tutte le responsabilità perché ne sono stata l'amministratore delegato, il presidente ed è quindi giusto che io risponda sulle cose di cui sono responsabile.

Ad oggi ovviamente rimango solo azionista di maggioranza, ma ho la certezza assoluta che i miei collaboratori (ex), che hanno lavorato con me da oltre venticinque anni, sapranno portarlo avanti bene e a lungo. Con il mio gruppo ho agito come avrebbe agito qualsiasi imprenditore che vive la crisi endemica di quel settore. Non ho avuto favoritismi, né li ho cercati. assunto invece iniziative per contrastare l'andamento del mercato e ho separato le due attività mediante la costituzione di un veicolo quotato in borsa per quanto riguarda l'attività editoriale. Qui avverto il dovere di una puntualizzazione. La società quotata, nella sua fase di ristrutturazione, ha fatto ricorso a prestiti obbligazionari convertibili, perfettamente legittimi e in linea con le direttive di Borsa Italiana e di Consob, da parte del fondo Negma; fondo che negli ultimi anni utilizza questo strumento non solo sulla piazza d'affari milanese, ma anche sulle piazze europee. A tal proposito, potete leggere l'articolo di "Milano Finanza" di pochi giorni fa, che al riguardo elenca le varie attività del gruppo Negma in tutta Europa; un fondo che opera come tanti altri fondi dello stesso genere, e posso citare il fondo ABO, il fondo Atlas, Nice & Green e tanti altri. Da settimane, però, si insinua che dietro il fondo in questione vi sarebbero presenze ignote. Ignota mi è invece la fonte di questa insinuazione. Come è nella sua abituale attività di fondo, il fondo Negma è venuto a cercare e a offrire il suo interesse per Visibilia SpA, quotata in borsa. Verificato che era un gruppo regolarmente attivo in molti Paesi europei e che in Italia aveva già fatto operazioni similari con altre società quotate - ad esempio con Blue Note e con Casta Diva - non abbiamo avuto motivo di non accettare il suo intervento. Quando poi un socio di minoranza, residente nelle Bahamas - di cui credo di aver detto tutto prima - ha avanzato proposte per noi irricevibili, lo abbiamo contestualmente diffidato tramite uno studio legale, che - sia detto per inciso - è l'unico intervento professionale, peraltro amichevole, dello studio legale La Russa nella vicenda della quale ci stiamo occupando. Quello che posso dirvi è che, per risanare le imprese, ho immesso tutta la liquidità di cui disponevo, per estinguere - come ho fatto - integralmente tutti i debiti, in primo luogo quelli fiscali. Ma questo non l'ha mai detto nessuno, pur essendo un fatto ampiamente noto, riconosciuto e documentato, sul quale tornerò in chiusura. Anche in questo caso va fugato ogni dubbio. Che l'intervento del fondo Negma anziché danni abbia portato vantaggi è pacifico. Al termine del processo e con l'ingresso di un nuovo socio di maggioranza, che a sua volta ha provveduto a completare l'operazione, il titolo ha guadagnato in borsa da gennaio oltre il 500 per cento e, dalla data della diffusione della trasmissione televisiva, ha guadagnato un altro 200 Per trasparenza vi dico, prima che succeda qualcos'altro, che non ho più alcuna partecipazione azionaria nella società in questione. Ma credo - lasciatemelo dire - di aver avuto il merito di aver creato le condizioni per questa situazione molto positiva per il mercato. Per fare un esempio, a fronte di tale risultato borsistico di Visibilia SpA, ci sono realtà editoriali quotate in borsa, che si sono quotidianamente occupate di me in questi giorni, le quali hanno perso invece oltre il 40 per cento del valore dal giorno della loro quotazione. All'interno di Visibilia SpA c'era una dipendente *part-time*, riguardo alla quale sono stata accusata giornalisticamente addirittura di truffa ai danni dello Stato, per aver dichiarato che era in cassa integrazione a zero ore, a sua insaputa, mentre la società avrebbe continuato a fruire delle sue prestazioni. In questo caso abbiamo dunque un lavoratore che riceve le buste paga, che indicano la sua collocazione in cassa integrazione, che dice però di non saperlo e nega di essere stato informato. Al di là di questa notazione, stiamo ai fatti. Di fronte alla contestazione tardiva della dipendente sulla cassa integrazione, pur ritenendo le sue affermazioni infondate e pur essendo io certa che quella dipendente non ha mai messo piede in Visibilia dalla sua entrata in cassa integrazione, la società ha preferito sanare la posizione, considerando la lavoratrice in servizio per tutto il periodo e pagando le relative retribuzioni, contribuzioni e ritenuti fiscali, senza che fosse pervenuta alcuna richiesta dagli enti preposti e molto prima della vicenda mediatica di cui oggi parliamo. Va aggiunto che nessuna questione relativa alla cassa integrazione è mai stata sollevata da qualche altro dipendente di Visibilia. Anche queste circostanze vengono totalmente taciute nella trasmissione, che ha preteso di lanciare una notizia bomba, ma che in realtà è una non notizia. Devo avviarmi alla conclusione e voglio chiudere con il quadro complessivo della situazione del gruppo di società della pubblicità e dell'editoria. Le società Visibilia sono attualmente quattro: capisco che è un po' complicato, perché si chiamano tutte Visibilia. C'è anche Visibilia SpA, che ormai è definitivamente uscita dal mio controllo. Alla fine del 2022, la procura della Repubblica di Milano ha proposto nei miei confronti, per tutte e quattro tali società, istanza di liquidazione giudiziale,

che non credo possa essere sospettata di favoritismi nei miei riguardi, ha ritirato le istanze proposte, dopo aver verificato la totale estinzione dei debiti. Con riguardo alla società tuttora operativa nel settore pubblicitario, la stessa procura della Repubblica ha già preso atto che tutti i debiti sono estinti e dunque ha chiesto al tribunale fallimentare di differire la definizione Con riguardo alla quarta società, non operativa, è in corso una procedura di risanamento, che prevede il completo soddisfacimento dei creditori. Nessun creditore si è opposto al risanamento proposto nei termini ormai trascorsi e quel giorno era il 28 giugno. Questo fa ritenere vicina la definizione auspicata. Credo di essere stata chiara al riguardo, ma c'è ancora un altro dato che rende il quadro più chiaro. Per la complessa operazione di risanamento - come ho detto prima - ho messo a disposizione il mio patrimonio. Consentitemi di dire che per tutto ciò mi sarei forse aspettata un plauso, perché sfido chiunque a indicarmi un numero cospicuo di persone che impegnano tutto il patrimonio per salvare le proprie aziende. Ho quindi cercato di illustrarvi tutto senza finzioni, senza nascondere alcunché. Per quanto invece riguarda l'addebito che è stato mosso alla mia persona per la vicenda del comparto Ki Group, ribadisco che non ho mai avuto poteri e soprattutto che, fino a quando ho ricoperto, senza deleghe, la carica di presidente di Ki Group, la società era in ottima salute. Gli appunti mossi a tale società negli anni 2022-23, veri o falsi, esulano da ogni mio possibile intervento, essendo già uscita da tutto, da ogni organo, e avendo mantenuto - questo sì - il 5 per cento della partecipazione. Per quanto riguarda Visibilia, fermo restando che mentre «Domani», ripreso stamattina da «la Repubblica» *online*, assumeva il contrario, non sono raggiunta ad ora da alcun avviso di reato e men che meno da alcun rinvio a giudizio, che - quello sì - consentirebbe di muovere critiche politiche al mio operato prima di un giudizio definitivo. Preciso che le quattro società di pubblicità ed editoria, in crisi come tutto il settore, sono state oggetto - come vi ho detto - della procura di Milano. L'istanza è stata poi ritirata dalla procura stessa per due delle quattro società; per la terza ho già verificato le condizioni per il ritiro, mentre per la quarta - per la quale conto di ottenere lo stesso provvedimento - vi comunico che l'*iter* è vicino alla conclusione. Cosa resta? Le immancabili note di colore sul mio abbigliamento, sul mio tenore di vita, sulle mie case, sulle mie amicizie, sui nomignoli che mi sono stati dati e, infine, financo su multe riferite erroneamente a me per per sosta vietata o circolazione in zone a traffico limitato, multe in realtà di competenza dell'Arma dei carabinieri, a cui ha dato in comodato gratuito una mia vettura per non gravare sulle auto di scorta di proprietà statale.

sono multe che devo pagare. Vi è una cosa che mi fa sorridere, perché guardate che ci vuole ben altro per spezzarmi, per cambiare il mio umore o per farmi diventare triste (sono una persona contenta di quello che ha nella vita,

quello che mi fa sorridere, per il mio ottimismo, il mio buon umore e forse la mia forza perché, come diceva mio padre, ottavo figlio di contadini, solo chi ruba nasconde io non ho nulla da nascondere), è che le critiche più feroci vengano da molti che in privato hanno tutto un altro atteggiamento nei miei confronti

Per il resto, se ho commesso errori, ho già pagato, animata da una sola, solida certezza: gli organi giudiziari italiani, a partire da quelli fallimentari, funzionano bene, al di là - lasciatemelo dire - dei tempi forse un po' troppo lunghi. Sì, Presidente. Alla fine sarà solo quella la verità, la verità che purtroppo coloro che oggi parlano e scrivono pagine intere non faranno sapere a nessuno.

Signor Presidente, colleghi, innanzitutto permettetemi di cominciare esprimendo sincero e convinto apprezzamento per la decisione del Ministro di informare il Parlamento. Non era un atto dovuto e necessario. È frutto della sua sensibilità istituzionale, un gesto di rispetto nei confronti del Parlamento, ma anche e soprattutto di tutti i cittadini italiani. La sua informativa prende spunto da un'inchiesta giornalistica, meritevole di rispetto, ma pur sempre un'inchiesta giornalistica. Faccio questa premessa perché è sulla distinzione tra i due piani, quello giornalistico e quello giudiziario, che si svilupperà il mio ragionamento. La nostra posizione, in piena coerenza con la nostra storia, che non è mai a corrente alternata, è nitida: siamo garantisti e il nostro non è un garantismo a senso unico. Anche per questo motivo, trovo inaccettabile ed allarmante che, come abbiamo letto oggi su una testata giornalistica, il «Domani», venga pubblicata la notizia, vera o falsa che sia, di un possibile coinvolgimento giudiziario del Ministro. È semplicemente inquietante che la persona interessata, un libero cittadino, un Ministro del Governo, lo apprenda dalla stampa: e potrebbe purtroppo capitare a qualsiasi cittadino italiano. Se così è, questo sarebbe un fatto gravissimo, che supererebbe la vicenda di cui stiamo parlando in quest'Aula. Ci torna alla mente la notizia dell'avviso di garanzia all'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi durante un *summit* sulla criminalità organizzata a Napoli nel 1994, notizia che venne anticipata da un importante quotidiano italiano. Una vicenda che, come tutti sappiamo, si concluse con l'assoluzione di Silvio Berlusconi. Le parole da lei pronunciate oggi, signor Ministro, fanno chiarezza. Da un lato, le rinnoviamo la nostra fiducia e, dall'altro, ci auguriamo che il suo intervento oggi contribuisca ad attenuare i toni dello scontro politico e a svelenire il clima che si sta creando su questa vicenda. Non possiamo pensare che il Parlamento si trasformi in un'aula giudiziaria, dove si consumino processi con tanto di sentenze che, evidentemente, avrebbero il sapore della strumentalizzazione politica. Lasciamo fuori da qui, cari colleghi, i ruoli e i contesti che appartengono, per loro natura, ad altri luoghi: le sedi giudiziarie. Dall'opposizione si sta scatenando una campagna contro il Governo, non su argomenti politici, ma su altre questioni, di ben altra rilevanza. Purtroppo, torna in scena l'uso politico della giustizia. Non è un caso che ormai, da quando questo Governo si è insediato, le minoranze si esercitino a chiedere, a turno ovviamente, le dimissioni di qualcuno. Abbiamo superato, se non sbaglio, la decina di richieste di dimissioni. Ormai ce n'è per tutti:

per questo motivo, le parole pronunciate qualche giorno fa dal senatore Matteo Renzi, che ha detto: io non attacco sulla Santanchè, ma preferisco attaccare su argomenti politici. Auspichiamo quindi che, una volta espletato questo passaggio, si possa tornare a discutere delle questioni che stanno davvero a cuore ai cittadini italiani: lavoro, sostegno alle imprese, sicurezza, sanità pubblica o politiche sociali.

Lasciamo questa tentazione a chi nell'opposizione si assumerà tale responsabilità. Noi della maggioranza stiamo dalla parte della legge e dunque, per definizione, esprimiamo da sempre massima fiducia nell'operato della magistratura. Per questo motivo, esprimiamo convintamente il nostro sostegno e rinnoviamo la nostra fiducia al ministro Santanchè.

alle sue dipendenze. Lei ha ammesso adesso che avete provveduto a sanare una situazione, quindi ha parzialmente ammesso che c'è stata una defezione da questo di vista. Le fosse vero che molti dipendenti sono stati licenziati e non hanno avuto il TFR. Anche su questo punto ha detto che non dipende e non spetta a lei, ma verranno pagati. Questa è un'ammissione del fatto che ci sono lavoratori e lavoratrici che nei processi di ristrutturazione delle sue aziende sono stati licenziati e non hanno ancora avuto il TFR. Questa è una seconda domanda a cui non ha risposto. In terzo luogo, le abbiamo chiesto e continuiamo a

SCN))*. Signora Ministra, la ringrazio per essere venuta qui oggi e per averci parlato come ha fatto. Le auguro davvero che quanto sta emergendo - ammesso che ci sia qualcosa che emergerà in questi giorni - non abbia un risvolto giudiziario e, se così fosse, le auguro di dimostrare di essere del tutto estranea ai fatti. Vorrei però ricordarle che situazioni di questo tipo sono state vissute frequentemente anche in passato nel nostro Paese e spesso riguardavano membri del Governo di tutti i colori. Ovviamente non abbiamo fatto una bella figura. Tutte le volte che un Ministro rischia di essere considerato uno che infrange le leggi viene meno l'immagine del nostro Paese. Io sono assolutamente dell'avviso che sia meglio che non succeda, per cui davvero le auguro di venirne fuori pulitissima, come lei ha detto poc'anzi. Mi consenta però qualche considerazione rispetto a quello che rappresenta un po' anche la sua persona e la sua figura di politico. Nell'immaginario del Paese lei rappresenta un tipo ideale di politico di centrodestra della seconda Repubblica, cioè quello che ha la concezione rispettabilissima e del tutto legittima che le imprese sono il volano del benessere, che vada deregolamentato quindi il mercato del lavoro, vadano diminuite le forme di controllo dello Stato e vada ridotta la tassazione, magari anche a costo di manomettere lo Stato sociale e di abolire il reddito di cittadinanza, di cui è sempre stata una fiera oppositrice. Ripeto che sono tutte cose assolutamente legittime, che rientrano nella dialettica democratica. Tuttavia il mio pensiero, leggendo quello che hanno scritto i giornali e dopo averla ascoltata ora, va ai tanti piccoli imprenditori che sono davvero la spina dorsale del Paese e che durante la pandemia hanno davvero dimostrato il valore sociale del fare impresa. Quindi, se tutto quello che è stato scritto anche in qualche piccola misura fosse parzialmente confermato, mi chiedo che cosa potrebbero pensare di questa vicenda quelli che hanno la villetta attaccata al capannone, quelli che vivono gomito a gomito con i propri operai o quelli che hanno rinunciato ai propri compensi per garantire gli stipendi e non licenziare nessuno. Mi chiedo che cosa ne potrebbero pensare quelli che perdono una parte della loro giornata a districarsi tra burocrazia e inefficienze del sistema, quelli cui le banche e il fisco non fanno sconti e che, se chiedono un prestito o hanno un debito verso un fornitore, passano notti insonni. Mi chiedo anche che cosa potrebbero pensarne i tanti ragazzi cui anche lei in questo tempo ha detto che non bisogna poltrire sul divano, quelli che vengono invitati a rimboccarsi le maniche e ad accettare lavori umili e precari anche quando la paga è sotto la soglia di accettabilità, perché tanto quello che conta è fare esperienza. Tutto questo mi fa venire in mente un celebre monologo di Alberto Sordi, che forse è il caso di avere sempre presente. Capisco allora, da un lato, il tono laconico da atto d'ufficio con cui la maggioranza ha preso le sue difese; al di là dei possibili risvolti giudiziari - su cui, lo ripeto, le auguro il meglio - questa sua vicenda ha dentro tanti elementi di criticità da essere oggettivamente fonte di imbarazzo per chi ha costruito le proprie fortune politiche sulla contrapposizione tra quelli che non hanno mai lavorato in vita loro e i cosiddetti uomini del fare. In questi giorni è stato detto che in altri Paesi per molto meno ci si dimette. Vede, signora Ministra, secondo la mia e la nostra concezione di etica, in considerazione dei suoi interessi economici, che non ha ritenuto di delegare a terzi al momento di diventare Ministra, lei non avrebbe neanche dovuto accettare l'incarico, perché nel farlo non sarebbe stata né la prima, né l'ultima e sarebbe stata solo una che di buon grado si fa carico dell'unico pegno richiesto a chi si trova nella condizione di privilegio di essere Ministra, cioè tenere rigorosamente separato l'interesse privato dell'imprenditore da quello pubblico che ogni Ministro è impegnato a perseguire. *(Applausi)*. Questo sì, sarebbe stato un vero atto politico,

Ministra, con quale metro di giudizio e con quale pietra di paragone dovremmo analizzare il suo discorso e la sua situazione oggi? Vede, signora Ministra, se dovessimo impiegare il metodo che era usuale nel suo partito e in quello della *Premier* dovremmo usare toni molto diversi. Desidero richiamare all'Assemblea quando, in condizioni analoghe, ci furono atteggiamenti diversi, anche da parte sua. Ricorderà senz'altro la vicenda dell'allora ministra Idem. Cito testualmente: "le dimissioni sarebbero un gesto significativo di rispetto delle istituzioni" (Giorgia Meloni); "fosse successo a noi, saremmo già state cacciate" (Daniela Garnero Santanchè). Ne approfitto, signor Presidente, per mandare a Federica Guidi un pensiero di vicinanza e di condoglianze in una giornata così dolorosa per lei.

Non c'è dubbio che la Boschi avrebbe dovuto dimettersi, perché nel caso Etruria" non è vittima di un linciaggio sociale, e avrebbe dovuto dimettersi molte volte in questi mesi" maggio e dicembre 2017). Fin qui il campionario delle dichiarazioni, a cui si potrebbe anche aggiungere quello delle casistiche.

ricorderà forse gli avvisi di garanzia di quella che venne definita mafia capitale e la richiesta di dimissioni al sindaco di Roma dell'epoca, non indagato, fatta da Fratelli d'Italia. Ricorderà forse il giugno del 2017, quando Giorgia Meloni chiese le dimissioni del ministro Lotti nel caso Consip, per il quale è stato assolto il generale DelSette; ricorderà forse il dicembre del 2017, quando Beppe Sala venne indagato per concorso in abuso d'ufficio (il reato che forse vi accingete a cancellare), per il quale voi chiedeste "dimissioni immediate". Ricorderà forse la vicenda di Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, indagata e poi prosciolta da ogni accusa, per la quale chiedeste e otteneste dimissioni immediate, che hanno cambiato il segno politico di quella Regione. Ricorderà senz'altro Bibbiano e Giorgia Meloni che andava a Reggio Emilia chiedendo le dimissioni di tutti gli amministratori del Partito Democratico e del centrosinistra.

Partendo anche da questa situazione, vogliamo sottrarci al ruolo intercambiabile del gioco delle parti, che ci porta ad essere garantisti quando governiamo e giustizialisti quando siamo l'opposizione? Noi sì, ci vogliamo sottrarre a questo gioco. Vogliamo emanciparci dalle caratteristiche di questa Seconda Repubblica, che ha trasformato i parlamentari da attori della politica a novelle *tricoteuse* intente ad assistere dalla prima fila alla decapitazione del politico di turno, in omaggio a un giacobinismo sfrenato. Noi sì, ci vogliamo sottrarre.

al Paese. Noi, infatti, distinguiamo tra la responsabilità politica e le vicende giudiziarie, anche se lei ci ha tenuto a rimarcare che ad ora non ha avuto procedimenti di natura giudiziaria. Qui però siamo a fare politica, quindi noi non chiediamo a voi le dimissioni come voi le avete chieste a noi. Noi oggi diciamo che ogni valutazione sul prosieguo della sua esperienza ministeriale è nelle sue mani e nelle mani del Presidente del Consiglio, che si assume la responsabilità politica e se c'è dell'altro, e può saperlo solo lei, tragga le naturali e necessarie conclusioni, perché la valutazione del tutto politica di questa vicenda e di questa decisione è tutta nelle sue mani. Grazie Forza Italia è e rimane il principale interprete del garantismo giuridico di questo Paese e non a pendolo e a seconda delle circostanze: non siamo garantisti per gli amici e manettari per gli avversari politici. Questo è il nostro DNA e ci vantiamo proprio di essere così. Per noi la bussola rimane sempre orientata sul principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, fissato dall'articolo 27 della Costituzione. Nel caso in esame la questione è posta sulla base solo - e lo sottolineo - di inchieste giornalistiche, informazioni e indiscrezioni di stampa. Detto questo, Presidente, la discussione si potrebbe anche chiudere qui. Per questo Forza Italia, e per essa la mia Capogruppo che siede qui al mio fianco, si era dichiarata fortemente contraria a questa informativa, richiesta dalle opposizioni o di parte delle opposizioni, che inevitabilmente rischia di trasformare quest'Aula in un'arena mediatica. Questo è il Parlamento, non un tribunale, né un ufficio di procura. *(Applausi)*. Non ci hanno insegnato niente tanti processi mediatici celebrati in Parlamento, a partire da quelli che hanno interessato Silvio Berlusconi e dall'informazione sull'avviso di garanzia che gli arrivò all'inizio della sua carriera politica, mentre presiedeva un vertice internazionale, che hanno interessato però tanti altri politici che poi nel tempo sono stati assolti, processi politici sommari, che hanno fatto tanto danno alle persone, risolti poi in tante bolle di sapone? Le dico questo, signora Ministra, perché abbiamo apprezzato le sue parole e i suoi chiarimenti. Ora mi consenta, Presidente, qualche considerazione in fatto e in diritto. Un primo dato: allo stato, la ministra Santanchè non è stata condannata da nessun tribunale e neppure rinviata a giudizio; nelle ultime ore, alcuni quotidiani hanno parlato di una fantomatica iscrizione nel registro degli indagati, che la signora Ministra ci ha appena spiegato sarebbe addirittura in un'inchiesta secretata, trapelata

Questa non è politica, ma barbarie, populismo giudiziario, giustizialismo manettaro. Presidente, se anche la Ministra fosse indagata, cosa cambierebbe? Attendiamo quanto meno che un giudice si pronunci. La senatrice Santanchè è venuta qui oggi non a parlare della sua attività di Ministro, ma della sua attività di imprenditrice. E trovo anche abbastanza surreale - se me lo consente - che sia dovuta venire a spiegarci le azioni, i soci e le obbligazioni convertibili, che sono cose del tutto estranee alla sua attività politica. Come tutti gli imprenditori, ha assunto un rischio d'impresa. Qui dentro tante volte celebriamo gli imprenditori, quelli che gettano il cuore oltre l'ostacolo, navigano in mare aperto e affrontano le insidie del mercato. Sappiamo tutti bene che il rischio d'impresa può far sì che le cose vadano bene - e noi lo auspichiamo che vadano bene, come ci auguriamo che a tutti gli imprenditori vadano bene - ma può anche succedere che vadano male

dei colleghi abbia oggi evidenziato nel suo intervento. La senatrice e ministra si sta adoperando con il massimo impegno per cercare di evitare il dissesto; lo ha già fatto e lo sta continuando a fare. È giunta al punto - lo dichiara oggi anche un giornale - di aver messo a disposizione delle procedure di liquidazione addirittura la sua casa di Milano. Questo è un gesto che le fa onore, Ministro: glielo voglio dire, perché la mette la mette in sintonia con tanti imprenditori che abbiamo visto in questi anni in difficoltà... Io le auguro sinceramente, Ministro, che quella casa non debba poi finire male, che le cose vadano meglio e che si possano risolvere, ma certamente volevo ribadirle, da parte mia, il massimo rispetto per gli sforzi e i sacrifici che sta facendo da questo punto di vista. Mi consenta un'ultima dichiarazione, Presidente. Chi ha voluto Chi ha voluto questa informativa cercava di trovare una maggioranza non compatta. Io credo che la visione che oggi tutti abbiamo qui dei Ministri schierati a fianco della ministra Santanchè ci dia invece il segno di una solidarietà forte, concreta e reale, che è quella che anche a nome di Forza Italia le voglio manifestare. Grazie ancora, Presidente, anche per la pazienza.

Santanchè, non continuo l'elenco fatto dal senatore Borghi, ma mi chiedo soltanto cosa sarebbe successo se su quel banco ci fosse stato un Ministro del MoVimento 5 Stelle e su questi ci fossero stati la ministra Santanchè e Fratelli d'Italia. Credo che non avremmo sentito gli stessi toni. Lei ha descritto, Ministra, la sua storia imprenditoriale vista dal suo cono d'osservazione. Leggendo bilanci di società, possiamo dire invece che forse è una storia un po' atipica, che lascia comunque una scia di debiti. Abbiamo ascoltato la sua esposizione, scritta probabilmente assieme ai suoi avvocati, però, vede, lei si dichiara estranea su molti fronti: ha citato il caso di Ki Group, dicendo che per tutto il 2022 lei non ci aveva nulla a che fare; fare; carta canta, però, e la carta è quella pubblicata sul sito del Senato. Faccio un breve ripasso: dal 2018 e fino certamente al 10 ottobre 2022, oltre a numerose partecipazioni societarie, nella dichiarazione che si rende al momento delle elezioni e che lei conferma di anno in anno ha dichiarato di essere amministratore unico di Visibilia, Biofood, Immobiliare Dani, D1 Partecipazioni, amministratore delegato di Visibilia Editore, presidente del consiglio di amministrazione di Bioera, che lei non ha citato nella sua relazione, e presidente del consiglio di amministrazione di Ki Group. Lei lo conferma fino al 10 ottobre: sta scritto agli atti del Senato. Quindi, evidentemente, anche nel 2022 era presidente di quel gruppo,

Qui non è in contestazione una fattispecie di reato. Questa è l'Aula del Senato della Repubblica e i reati si discuteranno casomai altrove e saremo contenti se lei riuscirà a dimostrare la sua estraneità ad ogni eventuale fattispecie di reato. Qui rileva una valutazione rispetto alla disciplina e all'onore con cui si esercitano incarichi

fanno parte della vita di ciascuno di noi, tanto più di un imprenditore, che assume e si accolla il rischio d'impresa. Ci sono però tanti modi di avere insuccesso, tanti modi di fallire e tanti modi di gestire la ricchezza e amministrare i soldi. Ricordo quando, in numerose trasmissioni televisive, attaccava quelli che chiamava i furbetti del reddito di cittadinanza. Una volta si è scagliata contro un padre di famiglia, un ex imprenditore percettore del reddito *(Applausi)*, dicendo che si doveva vergognare davanti ai propri figli. Non credo che sia lui a doversi vergognare: dovrebbe farlo farlo lei, per quelle parole. Non lo dico per demagogia, perché il reddito di cittadinanza era a disposizione di tutti, così come tante delle misure che lei ha detto di aver preso. Le sue società hanno avuto una grandissima capacità, quella di usare tutti gli ingenti fondi pubblici messi a disposizione delle imprese dal 2020. Ne faccio un rapido elenco, non esaustivo, perché tra il 2020 e il 2021 alla Ki Group sono stati concessi 1,38 milioni di euro di garanzia dello Stato (lo Stato siamo noi, quindi sono i nostri soldi), tramite Invitalia 2,7 milioni di euro di prestito garantito, 600.000 euro di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate e 740.000 euro di garanzie a Visibilia concessionaria e ha preso pure 2.000 euro a fondo perduto, che non mi sembra un valore particolarmente eccessivo, visto il suo tenore di vita. A questo quadro si aggiunge anche la cassa integrazione in deroga durante la pandemia, quella che lei diceva di dover anticipare ai suoi dipendenti, perché il Governo Conte non era in grado di erogarla, di cui però anche le sue imprese hanno beneficiato, anche se sembra che non tutti i suoi dipendenti ne fossero a conoscenza. Mentre lei in TV si sgolava tutti i giorni per attaccare il secondo Governo Conte, le sue società sfruttavano lecitamente *(Applausi)*, fino all'ultimo centesimo, ogni contributo pubblico, pagato anche dalle tasse dei dipendenti e di chi oggi ancora aspetta il TFR. A proposito, lei li ha citati poco, ma oggi ad assistere ai lavori dell'Assemblea ci sono delle persone: Ennio, Luca, Raffaella, Maria, Milena e Monica. Non so se le riconosce, ma sono suoi ex dipendenti, ai quali va il nostro applauso. il punto è il seguente: è questo il modello di impresa che portiamo in giro per il mondo, attraverso il suo incarico ministeriale? riteniamo che lei stia facendo un danno d'immagine enorme ai tanti, tantissimi imprenditori seri e capaci, che hanno bene a mente, soprattutto in questo momento, che cosa significhi la responsabilità sociale d'impresa. C'è un'altra sua dichiarazione che mi ha molto colpito in questi anni, che ha reso in una trasmissione televisiva in cui i bambini interrogavano i politici. Alla domanda di una bambina su cosa fosse il valore e il significato dei soldi, lei ha risposto: «Il denaro è l'unico vero strumento di libertà.

soprattutto se quel lusso e quella ricchezza sono il frutto del proprio lavoro e del proprio sacrificio quotidiano. Quello che non riteniamo accettabile è che il titolare di un incarico pubblico ostenti il proprio tenore di vita in modo plateale, avendo però costruito il proprio benessere economico anche sulle spalle degli altri. Lei oggi è in grado di guardare quei suoi *ex* dipendenti negli occhi? Non lo so. La presidente Meloni, com'è stato detto, in passato, anche se a corrente alternata, ha chiesto le dimissioni di alcuni Ministri per molto, molto meno. Lei oggi non ha convinto l'Assemblea e non ha convinto certamente noi; comunico che

perché questo lo troviamo un fatto molto preoccupante che dà la dimensione dello stato di salute in cui si trova la politica italiana in generale. Sostanzialmente, più passa il tempo e più la politica italiana conta sempre meno: questa è la riflessione che bisognerebbe fare seriamente. cui diceva che oggi non conta né la quantità, né tantomeno la qualità delle accuse. Oggi quello che conta è l'aspetto mediatico, il peso delle accuse mediatiche nei confronti delle persone. Si faceva riferimento in quell'articolo al passato, a si arrivò con la forza mediatica addirittura a far dimettere dei ministri - è stato ricordato prima da qualche intervento - che poi sono risultati perfettamente innocenti,

e dovremmo smettere di indebolirla giornalmente. Usiamo queste vicende per delegittimarci a vicenda mi riferisco alla famosa politica del garantismo a targhe

dei cittadini nei confronti del potere pubblico, in particolare di quello giudiziario. Tutto ciò dovrebbe farci capire che occorre essere garantisti, non solo con se stessi e non solo con i propri alleati o con i propri compagni di di Governo, ma anche e soprattutto con i propri avversari, perché solo in questo modo la politica potrà avere un domani.

le sue parole e devo dire che siamo rimasti impressionati; e non siamo gli unici, a giudicare, dal nervosismo che abbiamo percepito nei banchi del Governo e della maggioranza. Signor Presidente, lo voglio dire con chiarezza: il tema di questo dibattito non è il procedimento giudiziario per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio, di cui abbiamo letto su più organi di informazione, che sono reati gravi. Prendiamo atto, però, delle parole della ministra e, per noi, a differenza di tanti altri Gruppi che ho sentito parlare oggi, oggi, vale sempre il principio di presunzione di innocenza. *(Applausi)*. Noi oggi siamo il Senato della Repubblica, non un'aula di tribunale, ma abbiamo il dovere di discutere tra di noi su un tema, che non è un tema giudiziario, ma è una questione di opportunità politica e di credibilità delle istituzioni. Sono temi che richiedevano risposte chiare all'interrogazione che abbiamo presentato, alle domande rivolte dagli organi di informazione e da altri Gruppi parlamentari. Quelle risposte chiare noi non le abbiamo avute oggi dalla Ministra e, a questo punto, le chiederemo ai Ministri competenti. Chiederemo alla ministra Calderone dei lavoratori licenziati e rimasti senza stipendio e senza TFR. Chiederemo al ministro Urso delle ditte non pagate e messe in difficoltà. E chiederemo al ministro Giorgetti che fine hanno fatto i 2,7 milioni euro di soldi pubblici, di un prestito Invitalia, che non sono stati restituiti: perché questo è quello che emerge da quanto abbiamo letto negli organi di informazione. Signor Presidente, le dimissioni da Ministro sarebbero un gesto importante e significativo, un forte segnale di rispetto verso le istituzioni. Non sono parole mie: sono parole di Giorgia Meloni, pronunciate il 20 giugno

Meloni, che oggi non vedo tra i banchi del Governo, diceva: un atto di responsabilità, dopo quanto accaduto, è auspicabile. E negli anni, come hanno ricordato tanti colleghi, d'Italia e la stessa presidente Meloni non hanno risparmiato richieste di dimissioni e un atteggiamento intransigente nei confronti di tanti Ministri. Ecco, signor Presidente, è singolare questa conversione sulla via di Damasco della destra italiana. Intransigenti quando non erano i loro Ministri, oggi discettano di garanzie, di Stato di diritto, di attenzione: gli stessi che chiedevano le dimissioni per fatti molto meno gravi. *(Applausi)*. Stiamo ai fatti, signor Presidente. Nel caso in oggetto, quello che è emerso, e che non è stato chiarito dalle parole della Ministra, è una galleria di ombre, una galleria di brutture irrispettose nei confronti degli imprenditori che si fanno in quattro quotidianamente per pagare i loro dipendenti anche quando sono in difficoltà, per pagare i loro fornitori e per fare il loro dovere di responsabilità sociale.

la giustizia farà il suo corso, la ministra Garnero Santanchè, come prevedono le leggi di questo Paese, se dovesse essere coinvolta, si difenderà. Qui il tema è un altro, ma è un tema molto serio, è un grave problema di opportunità politica: può una Ministra di questo Paese, un membro del Governo della Repubblica avere una società che ha un debito nei confronti dello Stato italiano

*(Applausi)*. Può un Ministro che ha giurato di adempiere alla funzione pubblica che gli è stata affidata con disciplina e onore rimanere al suo posto di fronte a questa sequenza di fatti? Secondo noi no, non può rimanere al suo posto. «Cosa penso del caso Idem? Se fosse successo a una di noi del centrodestra, saremmo già state cacciate. Sono certa che Enrico Letta per il suo bene e per il bene del Governo la sostituirà». Ministra Santanchè, lo ha già detto il collega Borghi: queste sono le parole che lei ha pronunciato in un'intervista a «la Repubblica» il 24 giugno 2013. Oggi in quest'Aula noi le chiediamo di essere coerente con sé stessa, con quelle parole, con le parole che avete pronunciato in questi anni. Noi le chiediamo di rassegnare le dimissioni per il bene del Governo e per il bene delle istituzioni di questo Paese.

voglio dirlo subito nel modo più chiaro e deciso di cui sono capace: lei ha ancora più oggi che mai la piena fiducia mia e di tutti i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia, a nome del quale ho l'onore di intervenire. Voglio aggiungere che oltre alla nostra fiducia, da lei sempre ampiamente meritata, ha soprattutto tutta la nostra solidarietà per gli attacchi ignobili che ha dovuto sopportare da parte di alcuni organi di informazione, sedicenti, noti per la loro faziosità e molto più interessati e molto più interessati a infangare la sua immagine di quanto lo siano a raccontare la verità. Il caso del «Domani» che lei ha appena citato è emblematico. Ma quel che più dispiace di questa vicenda è dover constatare come alcune forze di opposizione, come già anche nel recente passato - vedi per tutti il caso Cospito si siano lasciate dettare la linea da certi organi di informazione, prendendo per oro colato notizie false, parziali o travisate, come il suo intervento, rispondendo a domande cui lei non era tenuta a rispondere in quest'Aula, ha ampiamente dimostrato. Le opposizioni sperano ancora una volta di mettere in difficoltà il Governo e di nascondere in questo modo la mancanza di idee e di linea politica in cui si dibattono, dimenticando persino la storia degli ultimi decenni, la quale insegna che questa strategia non solo non funziona, ma regolarmente si ritorce contro chi la pratica. Vorrei rispondere poi al collega Borghi e al collega Misiani. Le richieste di dimissioni da parte dell'opposizione sono assolutamente legittime, ci mancherebbe, lo facevamo noi e lo fate voi. lo fate ogni giorno, praticamente ormai si contano sulle dita delle mani i Ministri dei quali non avete chiesto le dimissioni per i motivi più disparati, sempre non inerenti all'esercizio del loro mandato

ai colleghi che mi hanno preceduto quanti casi conoscono di Ministri che sono stati costretti a venire a giustificarsi in un'Aula del Parlamento per fatti che non ineriscono al loro mandato.

È questo il vostro concetto di Stato di diritto e di democrazia parlamentare? Noi non lo condividiamo, cari colleghi.

sulle pagine pubbliche del Senato, perché la dichiarazione cui ha fatto riferimento, pensando di smentire il ministro Santanchè,

il senatore Patuanelli ha fatto riferimento alla disciplina e all'onore, con riguardo a fatti vecchi di anni,

Ormai siamo abituati da anni all'atteggiamento della sinistra. Ce lo ha insegnato «La fattoria degli animali» di George Orwell: per loro c'è sempre qualcuno più uguale degli altri; vogliono sempre essere più uguali degli altri. Peccato che la maggioranza degli italiani ha capito benissimo questo gioco e non vi segue più. Forse siete talmente disperati da farvi dettare la linea da giornali scandalistici, perché non avete più idee e non avete più prospettive politiche.

la ringrazio, per il suo tramite vorrei partecipare all'Assemblea la notizia della laurea di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna che questa mattina ha difeso la sua tesi in letterature moderne comparate post-coloniali una rara occasione di gioia per un uomo che da tre anni e mezzo vive l'incubo di una persecuzione assurda e feroce per la libertà delle sue idee in Egitto. Nel 2021 quest'Aula ha vissuto un momento legato a Zaki, con per il conferimento della cittadinanza onoraria alla presenza significativa della senatrice Segre, ma purtroppo tale mozione è rimasta un'aspirazione che non ha preso corpo. abbiamo chiesto al Governo di sostenere presso le autorità egiziane il diritto di Patrick di poter viaggiare, di poter lasciare il proprio Paese, ad esempio, per poter andare a Bologna a discutere la sua tesi ha consentito al regime egiziano di ignorare la richiesta di Zaki di vedere sterilizzato il suo divieto di viaggiare, cosicché questa mattina Patrick ha dovuto laurearsi a distanza, in collegamento e non in presenza. Presidente, il 18 luglio si terrà l'ennesima udienza del farsesco processo che lo vede imputato. Finora si è andati di rinvio in rinvio, con un'agonia personale che è agonia democratica, asfissia di diritto e di libertà, quella anche di muoversi fuori dall'Egitto. Peraltro tale permesso è stato accordato dalle autorità di quel Paese ad altri dissidenti sotto processo, ma non a Patrick, che pure è studente (oggi laureato con 110 e lode) dell'Università di Bologna. Ci sarebbe margine, spazio; sarebbe forse doveroso da parte del nostro Governo rappresentare all'autorità egiziana l'opportunità di revocare le limitazioni di spostamento. Non è stato ritenuto prioritario fino a oggi, come testimonia questa cerimonia da remoto, ma potrebbe, dovrebbe, può,

un intervento urgente, vocale, attivo del Governo italiano sull'Egitto. A noi qui oggi resta la gioia asprigna, la felicità mozza per un percorso che si chiude ed una traiettoria esistenziale che resta aperta, ma sotto schiaffo, ristretta, non libera, eppure viva, resistente, fiera, come la libertà che cerca e che merita, non come concessione, ma come diritto. Auguri Patrick! *(Applausi)*.

Uomo di grande intelligenza, perbene e di grande coraggio, purtroppo si è spento dopo una lunga malattia, ma neanche negli ultimi giorni ha smesso di lottare per quella che è stata la missione della sua vita, cioè portare a compimento la Torino-Lione, grazie anche alla sua determinazione e competenza ci siamo riusciti. Ormai nessuno potrà più tornare indietro da quest'opera e finalmente riusciremo a realizzarla. Per chi come me ha fatto e fa politica a Torino, Mario Virano è stato un maestro innanzitutto di stile, perché prima di tutto ha sempre pensato al bene pubblico, prima che gli interessi personali. Alla sua famiglia va ovviamente il cordoglio di Italia Viva e mi permetto di dire di tutti i torinesi e piemontesi che con lui perdono un grande maestro di stile, di competenza e di capacità. Mario, la terra ti sia lieve. Ti ringrazio per tutti gli insegnamenti che da sempre mi hai dato e per tutto il tempo che hai dedicato a me che ero una giovane appena arrivata in politica e col tempo sei stato orgoglioso dei miei successi, come un padre. Questo non lo dimenticherò mai e per questo ti mando un grande abbraccio. Mancherai a tutti noi.

dignitoso, estremamente duro nel difendere i diritti delle persone con disabilità, e dolcissimo nell'amicizia, la voglia di confidarsi e farsi farsi conoscere, nonostante si sentisse solo, anche se in una solitudine affollata considerate tutte le persone che nel dipartimento condividevano con lui la sfida, anche condivisa, di dare più dignità, libertà e parola alle persone con disabilità. Lui ne aveva una pesante, che portava con onore e dignità, appunto. Noi

in ogni modo, ai lavori della Camera alta per portare in alto i diritti delle persone con disabilità. Alessandro, tu sei con noi, rimarrai con noi e sarai per noi un esempio costante. Grazie, un bacio.